che può trovare spazio adeguato soltanto nel programma di una forza politica nazionale qual è il PdL e nel Governo della Repubblica italiana. Infatti, il presidente Berlusconi ben ha considerato questo aspetto sostenendo che il Mezzogiorno d'Italia è una questione che il Governo nel suo complesso - e, aggiungo, un grande partito nazionale nel suo complesso come il PdL - deve affrontare. anche su questo piano, rispettosamente ma convintamente, non sono favorevole a uscite o anche a formazioni estemporanee. Mi sembra che il problema del Mezzogiorno, che è di grande rilevanza, debba trovare posto debba trovare posto nell'agenda del PdL e del Governo come un grande problema nazionale. Questo credo sia fondamentale. Ci dividiamo naturalmente su tali questioni ma credo che la

polemica passi anche ad essere un po' demagogica non mi convince, perché qui parliamo delle agevolazioni previdenziali per l'agricoltura, in particolare per quella del Mezzogiorno. Devo ricordare che questo Governo,

prima istituito e poi prorogato le agevolazioni previdenziali per l'agricoltura, in particolare per i territori particolarmente svantaggiati, che sono quasi quasi totalmente nel Mezzogiorno d'Italia. Noi cioè abbiamo operato come un Parlamento ed un Governo devono fare, senza toni polemici, ma con norme, con provvedimenti che stanno attribuendo all'agricoltura il contributo che ci si prefiggeva

Ripeto, si può dire che non è stato fatto tutto, ma a questo punto potrei argomentare altro. E comunque questo è stato fatto e non si può dimenticarlo solo per foga polemica.

il modo di affrontare i problemi dell'agricoltura. Non bisogna porre veti o criticare ciò che fa l'altro, ma si devono unire le ragioni vere dell'uno e dell'altro e venire incontro ai problemi complessivi di un comparto importantissimo come l'agricoltura,

ha fatto il nostro Governo, così ha fatto la nostra maggioranza.

ennesima richiesta, preghiamo i colleghi senatori e il Governo di

che i Sottosegretari presenti nel momento in cui abbiamo dibattuto la conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2009hanno sempre detto che negli anni successivi si sarebbero trovate le risorse

il Governo ha visto approvare in Aula un ordine del giorno all'unanimità. Il ministro Tremonti ha allora detto, sulla questione del ristoro delle imposte sospese che ridecorreranno dal 1° gennaio, che con un'ordinanza si provvederà a modificare una legge.

il decreto-legge sull'Abruzzo

È la legge che prevede la possibilità, con le ordinanze, di disporre sospensioni. Quindi, con un'ordinanza si può modificare l'ordinanza vigente.

chiaramente insostenibile (perché non occorre essere scienziati del diritto per comprendere che le ordinanze di protezione civile si fanno sulla materia propria della protezione civile e non su disposizioni di carattere finanziario fissate per legge), a conferma della convinzione con la quale egli ha esposto la sua tesi, risulta non abbia partecipato al voto, evidentemente imbarazzato del voto che avrebbe dovuto esprimere per vincolo di maggioranza. Le chiedo, senatore Pastore, se questo corrisponde al vero e se anche gli altri colleghi abruzzesi abbiano o meno partecipato al voto (mi riferisco al senatore Tancredi, al senatore Di Stefano e al senatore Piccone), perché qui siamo in presenza di un fatto

nonostante stamattina sia stato molto ben argomentato in alcuni interventi il rapporto tra questo Governo e il Mezzogiorno. Perché non condivido l'impostazione e la formulazione della collega Poli Bortone? Perché quello che non si dice è che si vorrebbe un processo alle intenzioni filoleghiste di rappresentanti del Governo come i ministri Tremonti e Sacconi; si direbbe che è stato questo giocare a nascondino con i fondi del FAS a produrre ciò che il sociologo De Rita ha definito il "movimentismo meridionalistico" di questi mesi. In realtà, quali che siano le intenzioni di Ministri come Tremonti e Sacconi, speravo che tanto da parte della collega Finocchiaro, quanto da parte della collega Poli Bortone ci fosse la capacità di comprendere che la questione meridionale è scomparsa dall'agenda politica nazionale non per il leghismo, che è vicenda che risale alla fine degli anni '80, ma per l'istituzione delle Regioni, che è degli anni '70.

possibile discernere chi cofinanzia che cosa? Tanto più che il riferimento costituzionale molto pungente della collega Poli Bortone riguarda una riforma della Costituzione con cui sono

quella politica delle infrastrutture che ha consentito, invece, se non l'industrializzazione, la industrializzabilità del Mezzogiorno negli anni '50 e '60. Ho quindi la sensazione che ci sia una sorta di omertà regionalistica in queste formulazioni formulazioni e una sorta di pregiudiziale processuale nei confronti dei membri di questo Esecutivo. Di qui il mio voto contrario a questo emendamento.

A questo proposito è opportuno ricordare che nel nostro programma elettorale è scritto: (...)». Ora mi domando se in un Documento di programmazione economico-finanziaria si possa parlare di un programma elettorale non si sa bene di chi, forse di un Governo che ancora non c'era, di una forza politica, di tutta la coalizione. Forse la confusione dei piani ci aiuta a comprendere anche perché su questo emendamento, apparentemente in linea con i provvedimenti già approvati, questa maggioranza si esprima in maniera contraria.

come inutile. Però anche un rito inutile può riservare pezzi di verità. È stato per me un elemento di ulteriore rafforzamento nella giustezza della nostra impostazione cogliere alcuni voti di astensione tra le file del PdL sugli emendamenti

il dibattito su questo DPEF in qualche modo è stato in gran parte riservato alla materia dello sviluppo del Sud, di cui il Governo non si è occupato. Noi comunque questo rito l'abbiamo rispettato. Abbiamo pesato il DPEF e ne abbiamo valutato i contenuti. L'abbiamo poi ritenuto insoddisfacente, perché abbiamo ritenuto insoddisfacente, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, come lei sa bene, l'azione del Governo nei confronti del Mezzogiorno.

ritenuto insoddisfacente l'azione del Governo rispetto al programma elettorale. Al punto 5, signora Presidente ... Tante volte sento la Presidenza che raccomanda ai colleghi un po' di tranquillità quando parlano altri senatori. Potrei per una volta ottenere anch'io...

l'insoddisfazione del Movimento per le Autonomie per l'azione del Governo è legata al mancato rispetto del punto 5 del programma della coalizione, che recita: «Noi «Noi vogliamo un'Italia che finalmente superi, attraverso un impegno straordinario, il drammatico divario tra Nord e Sud, realizzando una politica che valorizzi la responsabilità dei territori e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese». Evito di leggere gli elementi che specificano questa asserzione di principio perché sarebbe la sagra delle incompiute o delle mai avviate. di questo nostro giudizio, da cui deriva una scelta politica precisa che riguarda i rapporti dentro la maggioranza di Governo, è che da questo momento in poi noi, come come Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud (denominazione che rende chiara la ragione del nostro impegno a fianco del Governo), valuteremo tutti gli atti del Governo in ragione della coerenza con questo principio programmatico della coalizione. E siccome abbiamo ritenuto che questo provvedimento non contiene le scelte strategiche che si fanno carico del recupero del divario tra Nord e Sud, noi non possiamo condividerlo. Il vice

avuto questo accento critico. Ma come faccio a non essere critico rispetto a un giudizio così dettagliato su tutte le inadempienze del Governo rispetto alla responsabilità che ha verso i territori meridionali? Aggiungo una cosa che notavo questa mattina rileggendo alcuni appunti sul DPEF. Dopo 15 anni dal 1994, anno in cui possiamo iscrivere l'inizio della mitica seconda Repubblica, il debito pubblico italiano è ritornato agli stessi livelli. La seconda Repubblica e tutte le sue politiche di controllo della finanza pubblica, di rigore e di

negli ultimi 11 anni (c'è quindi una certa contestualità temporale), ha perduto 700.000 persone emigrate (di cui 122.000 soltanto nel 2008) da Campania, Puglia e Sicilia. Dal Sud parte il 38 per cento dei laureati con il massimo dei voti. Il Mezzogiorno si è trasformato sempre più in «un'area periferica da cui si continua ad emigrare, dove crescono gli anziani ma non arrivano gli stranieri, dove esistono le realtà economiche eccellenti ma non si trasformano in sistema», anche per insormontabili difficoltà di accesso al credito che penalizza le forze sane e propulsive. Tra il 1990 e il 2001 abbiamo assistito al progressivo smantellamento del sistema creditizio meridionale, che ha visto diminuire del 46 per cento il numero delle banche dedicate. L'Italia è sempre più divisa in due: le dinamiche negative in termini occupazionali che agiscono in aree dove lavora solo il 44 per cento della popolazione in età da lavoro e dove le donne che lavorano sono meno del 30 costituiscono una situazione di potenziale emergenza assolutamente trascurata dal DPEF. Perché le dico questo, vice ministro Vegas? Perché questa mattina lei riteneva che i nostri accenti critici fossero ingiustificati rispetto al tanto che il Governo ha fatto. Il Governo si è ascritto come merito l'intervento per l'emergenza dei rifiuti in Campania e quello per il terremoto in Abruzzo. Lei mi vorrà consentire che io spero che non tutto il Mezzogiorno si precipiti in emergenze drammatiche come quella dei rifiuti in Campania o un terremoto per poter meritare l'attenzione del Governo! Non le pare già sufficientemente grave la condizione sociale ed economica del Sud perché questo Governo cominci a intervenire con strumenti che sono la semplice

che doveva consentire un intervento aggiuntivo rispetto all'intervento ordinario dello Stato che vale per tutto il territorio. Esso è però stato trasformato nel tempo in un intervento sostitutivo, per esempio rispetto alle grandi imprese pubbliche nazionali, come ANAS e Ferrovie,

non posso sostenere questo documento. Allo stesso modo, non posso considerare soddisfacente la formulazione generica introdotta per riconfermare un generico impegno sulla fiscalità di vantaggio. non vogliamo un trasferimento brutale di spesa pubblica da disperdere in mille rivoli, secondo gli antichi riti meridionali delle clientele, di cui dovremo discutere, perché le risorse dei fondi FAS, che sono state destinate destinate altrove, non erano di competenza delle Regioni meridionali e non erano né oggetto di programmazione, né oggetto di spesa delle amministrazioni periferiche: erano fondi di competenza dello Stato che devono essere programmati e spesi dallo Stato. ricordare che sul credito d'imposta automatico in un solo mese vi sono 23.000 richieste di finanziamento che esauriscono gli stanziamenti dal 2007 al 2013, e per il 2009 non vi è più un euro per il credito d'imposta automatico, meccanismo non di spesa pubblica, ma di incentivo allo sviluppo. Ecco, senatore Viespoli, lei ha scritto un articolo eccellente, pubblicato oggi sul quotidiano «Il Secolo d'Italia», in cui rilancia la fiscalità di vantaggio.

Questa formula - «valutare la possibilità» - per noi si è esaurita. Vogliamo scelte precise che impegnino il Governo a negoziare con l'Unione europea l'introduzione della fiscalità di vantaggio come strumento di incentivazione allo sviluppo. Per questa ragione, noi non voteremo la proposta di risoluzione Gasparri,

Signora Presidente, devo innanzitutto fare una considerazione di carattere preliminare che riguarda il Documento di programmazione economico-finanziaria. Il ministro Tremonti questa mattina, molto opportunamente, ha ricordato che dopo la riforma della contabilità pubblica, approvata quasi all'unanimità dal Parlamento,

elegante presentare proposte emendative ad un atto che non avrà alcun effetto per il futuro o quantomeno, al di là dell'attività di indirizzo politico, cambiate le regole di finanza pubblica e quindi anche i meccanismi...

cambiati i meccanismi di approvazione del bilancio dello Stato e dei documenti di programmazione,

Emendare cioè un atto che già nasce morto sembrava quasi infierire su un cadavere (mi si passi la metafora poco elegante). Devo dire che oggi il Governo e il Ministro hanno fornito una serie di elementi particolarmente istruttivi, che confermano

Quando questi dati sono stati resi pubblici e discussi in Italia ed in Europa, il Presidente del Consiglio ha definito catastrofisti questi organismi internazionali qualificati qualificati e anche gli organi di stampa che ne hanno parlato, perché rei di essere asserviti a qualche piccolo o grande complotto. Il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato per il 2010 (e basta) il il 15 luglio scorso stima la crescita economica del nostro Paese a meno 5,2 per cento più 0,5 per cento nel 2010. Io non so se queste sono previsioni catastrofiche, ma certamente sono peggiori di quelle stimate in sede europea ed internazionale. Delle due l'una, quindi: o siamo tutti vittima di una congiura internazionale, e non mi pare, oppure si è voluto nascondere agli italiani lo stato di criticità dei nostri conti pubblici. È evidente che i conti pubblici vanno male, perché la recessione determina il calo delle entrate e la crescita della spesa pubblica. Tra il 2008 e il 2009 l'indebitamento della pubblica amministrazione peggiora di 40 miliardi, passando da 40 a 80 miliardi, di cui 30 di incremento della spesa e 10 miliardi di minori entrate. Ora, è chiaro che questi dati non possono consentire di affidare alla buona fortuna l'andamento dei conti pubblici e la gestione delle entrate, come ci è parso di capire dall'intervento svolto dal ministro Tremonti in quest'Aula stamattina, in cui egli molto opportunamente ha chiarito opportunamente ha chiarito che il bilancio dello Stato in Italia è migliore rispetto al resto d'Europa e che c'è un *trend* che ci fa sperare che in futuro continuerà ad essere così. Sinceramente, con una decrescita del 5 per cento rispetto al prodotto interno lordo, questa previsione ha bisogno, secondo me, di essere assistita da un viaggio da Padre Pio! ricordavo, ha detto che questo sarà l'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria e che dal prossimo anno si passerà alla Decisione di finanza pubblica. Noi ce l'auguriamo, perché credo che dopo un anno di governo sia arrivato il momento di prendere qualche decisione vera ed importante nell'interesse del Paese. Infatti, signora Presidente, l'obiettivo che vi eravate prefissati di ridurre il costo complessivo dello Stato tagliando la spesa pubblica con una media del 3 per cento annuo è fallito. Se confrontiamo i dati del Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso anno e di quello presentato quest'anno, vediamo che nel DPEF, in valore assoluto, le spese dello Stato passano da 535 miliardi di euro dello scorso anno a 547 miliardi di euro di quest'anno. Esse quindi sono aumentate sia in termini di incidenza sul prodotto interno lordo che in valore assoluto. assoluto. Ancor più grave, cari colleghi, è che è cresciuta la spesa corrente ed è diminuita la spesa per investimenti, mentre nei periodi di crisi deve avvenire l'esatto opposto per garantire una efficace strategia di uscita - così parliamo in italiano, come dice il Ministro - dalla crisi. Le spese per investimenti passano infatti da 63 miliardi di euro a 55 miliardi di euro, mentre le spese correnti passano da 472 miliardi di euro a 492 miliardi di euro. L'aumento della spesa corrente, inoltre, non va a vantaggio né della famiglia italiana né delle fasce più deboli e a rischio di povertà sempre più presenti nel nostro Paese. Pensiamo ai tagli lineari nel settore dell'istruzione e degli enti locali. Sul terreno della riqualificazione della spesa pubblica non vi sono, inoltre, segnali positivi in controtendenza, ma ci si limita ad annunci e a norme che ostentano principi di efficienza ed economicità (assolutamente condivisibili) ai quali non segue mai alcuna pratica e positiva attuazione. Questo stato di cose determina solo ed esclusivamente un aumento del debito pubblico che non solo vulnera ogni strategia positiva di uscita dalla crisi, ma ipoteca il futuro dei nostri figli, condannandoli a pagare le tasse non per organizzare al meglio lo sviluppo del Paese, ma per tappare le falle create ed aggravate da noi. Stamattina su "Il Corriere della sera" Gian Antonio Stella citava il caso del commissariamento della Regione Calabria con riferimento alle spese sanitarie. È chiaro - lo dico senza alcuna polemica - che, se l'idea del risanamento passa attraverso la trasformazione dei governatori inadempienti in commissari risanatori, non si non si andrà da nessuna parte. Lo dico senza polemica politica, ma proprio perché oggi il problema è la crisi di sistema, cioè l'incapacità del sistema di governo dei territori, con questo pseudofederalismo, di dare risposte che non siano in termini di aumento della spesa pubblica e di aumento indiscriminato del prelievo e della pressione fiscale. Questa è l'operazione che avete fatto, e gli effetti nefasti del federalismo fiscale li vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quando avremo la possibilità di leggere il primo decreto attuativo della riforma federale. Non vi è stata in quest'anno alcuna manovra economica che abbia realmente affondato il bisturi nella spirale negativa nella quale ci troviamo. Si è deciso in altri termini di non decidere. E anche la manovra d'estate che esamineremo da domani non avrà alcun impatto netto sui saldi di finanza pubblica. Anzi, è l'ennesimo pasticcio istituzionale che vi costringerà prevedibilmente ad adottare un decreto-legge correttivo.

a sostegno dell'economia messi in atto dal Governo fino ad ora è stata di soli 3 miliardi di euro. Noi diciamo da un anno, in occasione di ogni provvedimento economico proposto dal Governo, che non è più possibile aggredire la crisi con manovre meramente correttive dei conti pubblici o, peggio ancora, con manovre che partono con lo scopo di aggredire le cause sociali ed economiche della crisi e che restano poi lettera morta. Non bastano più gli annunci buoni solo a far mutare l'atteggiamento psicologico dei consumatori italiani. L'ottimismo è, infatti, un elemento indispensabile di ogni disegno macro e microeconomico, ma da solo non basta. Occorre una chiara, coraggiosa e determinata azione riformatrice, a partire dalle pensioni, perché la spesa pensionistica - a causa della recessione - crescerà di più di un punto percentuale nel 2009, passando dal 14,2 per cento del 2008 Ciò che il Governo propone è l'equiparazione della età pensionabile tra uomo e donna nel pubblico impiego, assolutamente irrilevante sul riequilibrio dei conti previdenziali, ed una norma tendenziale sul riequilibrio della età pensionabile a partire dal 2015, quando cioè questo Governo non sarà più in carica. Non voglio citare qui le liberalizzazioni, ma voglio solo fare una considerazione sulla famiglia italiana, unico vero ammortizzatore sociale efficace nel nostro Paese, al Nord e al Sud. Credo che oggi l'unica vera riforma sia quella di cominciare ad introdurre progressivamente il quoziente familiare per rendere equa la tassazione nei confronti delle famiglie monoreddito, di quelle con più figli, di quelle con genitori a carico e di quelle con figli o genitori a carico non autosufficienti. Senza tale riforma non vi può essere né crescita di consumi, né della produzione. Signora Presidente, credo che altri siano i temi di cui dovrebbe occuparsi il Documento di programmazione economico-finanziaria, che sono invece messi nel cassetto perché la verità è che non ci sono

però, quando tirare a campare significa tirare le cuoia, credo occorra cambiare ragionevolmente e velocemente rotta, anche rispetto alle politiche del Mezzogiorno. Mezzogiorno. Su questo tema - e già tanti colleghi sono intervenuti in maniera molto autorevole rispetto a quello che posso dire io - credo che a settembre avremo la possibilità, se il calendario dei lavori ce lo consentirà, di svolgere un dibattito. Mi permetto Mi permetto però di fare solo una considerazione, e la voglio fare senza polemica nei confronti non solo dei colleghi della maggioranza, ma anche di quelli dell'opposizione che hanno votato il federalismo fiscale. Dalle nostre parti si dice che dopo che hanno rubato a Santa Chiara è inutile mettere le catene. L'operazione FAS, l'operazione conti pubblici, le leggi finanziarie e così via partono tutte dalla riforma del federalismo fiscale, che è la madre di tutti i problemi e della secessione economica e sociale di questo Paese. Da lì bisogna partire. E a questo riguardo vorrei dire a tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti che è inutile che parliamo di conferenze stampa e quant'altro. L'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale prevede già la cabina di regia, quindi non affannatevi e non affanniamoci; ci sono quattro Ministri Bossi, Tremonti, Calderoli e Fitto - chiamati a sostituire il CIPE e tutti gli strumenti di programmazione economica e finanziaria e che devono (anzi avrebbero già dovuto farlo, perché la legge è in vigore) programmare il fabbisogno infrastrutturale del nostro Paese. Quindi, di che cosa vogliamo parlare? È da lì che partono i guai e i guasti del nostro sistema e del nostro Mezzogiorno, dei quali abbiamo ancora visto solo l'antipasto.

c'è un calo dell'occupazione e della produzione anche nella parte imprenditorialmente più avanzata del Paese, che ha bisogno di assistenza, di quel tanto vituperato assistenzialismo di cui poi parlate nei confronti del Meridione d'Italia. Non ci stiamo lamentando, perché la politica del nostro Paese deve essere una e deve riguardare tutti i territori. Oggi avete bisogno, perché le vostre aziende sono in crisi, del sostegno della cassa integrazione ed è giusto che così si faccia, ma alimentare una guerra tra territori in questi termini è sbagliato perché non ci porterà da nessuna parte. Questo Documento di programmazione economica e finanziaria è ipocrita e non serve al bene del Paese.

abbiamo visto nella discussione che il DPEF che quest'anno siamo stati chiamati ad esaminare, con il suo elenco di dichiarazioni vuote, di risposte truccate, di misure inadeguate e tardive rispetto alla drammaticità dei problemi che vivono le famiglie e le imprese del nostro Paese, è un provvedimento svuotato di qualunque significato. Il primo a rendersene conto e a dichiararlo pubblicamente alla stampa (devo dire con una encomiabile quanto mai rara virtù di sincerità) è stato lo stesso Capo del Governo, quando ha dichiarato che nel DPEF non c'è niente di nuovo, non ci sono novità rispetto alla finanziaria triennale della scorsa estate. Andava bene prima e andrà bene anche di qui in avanti. Per noi non è così. In un anno dalla manovra estiva del giugno 2008 purtroppo sono cambiate - ed è peccato che il Presidente del Consiglio non se ne sia accorto - molte cose in Italia:

e poi scendendo, scendendo sempre più, sino al crollo attuale di oltre 5 punti percentuali del PIL, con un pesante aumento del debito e una disoccupazione stimata a due cifre. due cifre. Questa disoccupazione sta creando una dismisura di disuguaglianze mai sperimentata prima nel nostro Paese, non solo in termini di quantità, perché le cifre non danno il giusto senso delle persone in carne e ossa che perdono il posto di lavoro, ma anche di dignità della vita, che investe ormai masse di cittadini, superando i livelli di guardia. Con questo DPEF abbiamo l'obbligo di capire e di farci capire, senza la tragedia dei catastrofismi (certo, non da parte dell'Italia dei Valori), ma anche senza addolcire con ottimismi di facciata. Vedete, e lo dico ai rappresentanti del Governo, ci sono vari modi per essere, pur nella difficile congiuntura, ottimisti: c'è l'ottimismo dei tecnici, che si accontentano di guardare al rallentamento del ritmo di caduta dell'economia, concentrando la propria attenzione sugli indici premonitori e anticipatori; c'è poi l'ottimismo consolatorio di chi dice che in fondo nella nostra situazione poteva andare peggio; infine, c'è l'ottimismo che è segno di improvvisazione. Quest'ultimo è quello scelto dal Governo in carica. Il DPEF per noi certifica che questo Governo ha deciso di continuare per il momento a restare fermo. Nessuna riforma, in tutto solo 3 miliardi mobilizzati per sostenere l'economia nel mezzo della crisi peggiore del dopoguerra. I conti vanno male, perché calano fortemente le entrate e la spesa corrente cresce sempre e comunque. Ancora una volta si rinvia qualsiasi intervento o addirittura qualsiasi proposta di intervento sulla previdenza a quando il Governo non sarà più in carica, dal 2013 in poi. E lo stesso provvedimento sull'età della pensione per le donne nel pubblico impiego porterà a risparmi risibili. La ciliegina sulla torta è che si spaccia lo scudo fiscale come un provvedimento analogo a quello del Governo Obama. È cosa ben diversa, ditelo al ministro Tremonti: in Italia rimane l'anonimato sugli esportatori di capitali, in America c'è la *disclosure*; qui si paga una vantaggiosa sanatoria, là si pagano le imposte base. Eppure, il ministro Tremonti, che aveva promesso di non fare nuovi condoni, in spregio alla lotta senza quartiere all'evasione e ai paradisi fiscali propugnata nei *global legal standards*, offre un altro ennesimo regalo a chi non paga le tasse. Tuttavia, signor Vice Ministro, il vero giudizio politico sul DPEF non viene dato dai banchi dell'opposizione e dai tanti interventi, pur autorevoli e di spessore, che hanno dato contributi e suggerimenti. suggerimenti. Dopo 56 pagine di DPEF, tre allegati e un collegato al DPEF adottato soltanto pochi giorni fa, in cui il Governo si premura di spiegare la sua intenzione di continuare questa logica di prudenza fiscale e la sua prospettiva di guardare al dopo crisi nell'ottica di una riforma istituzionale dello Stato, per trasformare - come ci è stato detto - una crisi in un'opportunità, il vero giudizio di chi, dopo tutte queste belle parole, non si sente rassicurato da questi impegni del Governo e non crede nell'intuizione geniale di Tremonti (che ha avuto l'abilità di inventarsi il grande calderone finanziario dei fondi FAS, con il quale ha saputo alimentare di tutto e di più, dal terremoto dell'Aquila all'azzeramento dell'ICI dal risarcimento per gli obbligazionisti Alitalia al G8, dai fondi di garanzia per le piccole e medie imprese alla banda larga) proviene dagli stessi Ministri del quarto Governo Berlusconi, che sono andati all'arrembaggio. Stefania Prestigiacomo chiede 3 miliardi per i suoi progetti, Claudio Scajola ne chiede 2,8, Maria Stella Gelmini è solo al terzo posto di questa classifica con una richiesta di poco inferiore al miliardo e mezzo.Ci sono 700 milioni per il ministro Zaia; 600 milioni sono stati richiesti dal ministro Bondi, 330 dal ministro Brunetta e 150 dal ministro Maroni, con un'evidente schizofrenia tra i temi sventolati e la traduzione esattamente contraria, contrapposta e contraddittoria rispetto a quanto ritroviamo nel DPEF. C'è un altro limite in questa manovra, ed è il fatto che essa poggia su misure le cui modalità di attuazione non sono definite, per cui sono eventuali, incerte, future e di dubbia coerenza finanziaria. Di tutto questo, signor Vice Ministro, si sono accorte le Regioni, che sono partite all'attacco su sanità e fondi FAS: fino ad oggi abbiamo assistito ad un uso strumentale - stile bancomat delle risorse di questi ultimi, destinate allo sviluppo, mentre ancora non c'è certezza sulla liquidità di quelle già programmate e assegnate alle Regioni nel 2007.

e chi immagina un'ulteriore centralizzazione della programmazione non solo compie un errore di prospettiva, ma va in direzione opposta ai proclami del federalismo. Sulla sanità poi si sta giocando tra Governo e Regioni una partita difficilissima, anche perché quei 7 miliardi in più che tutti i governatori reclamano dal prossimo anno si stanno praticamente trasformando in una missione impossibile. E non va meglio per le infrastrutture: ho ascoltato in discussione un accorato intervento di un senatore del PdL della Sardegna, il quale, nell'Allegato alle infrastrutture, ha trovato per la sua Regione 19 milioni di euro e pensava che fosse un errore tecnico. Ci dispiace disilluderlo, ma non si tratta di un errore tecnico: l'articolazione negli anni della spesa per le grandi opere è inevitabile, lo sappiamo;

Un esempio? Gli 800 milioni stanziati per il MOSE di Venezia saranno spesi solo per un decimo (80 milioni) quest'anno, nonostante l'opera sia già in piena realizzazione. Un altro esempio? Il terzo valico di Genova riceverà quest'anno 500 milioni, un decimo del fabbisogno, e un ritmo di spesa tale da consentire la realizzazione dell'opera in trent'anni.

«meno male che Silvio c'è»: il Presidente del Consiglio si intesta subito il piano per il Sud, anzi, il piano Berlusconi, come ha detto chiaramente al Consiglio dei ministri; ci sarà cioè un piano Berlusconi per lo sviluppo del Mezzogiorno. Dopo il fallimento della Banca del Sud (che non sappiamo che fine abbia fatto), le prove per costruire il Partito del Sud e le tensioni ormai esplose nel Governo sulla ripartizione dei fondi FAS, il Capo del Governo cerca di correre ai ripari, tardivamente e

giro. In conclusione, è mai possibile che per noi dell'Italia dei Valori in questo DPEF non ci sia nulla di buono? Devo ammettere che resta interessante la posizione del ministro Sacconi sul *welfare* dei giovani, quando - bontà sua - dichiara la crisi economica può essere per i giovani una frustata salutare e un incoraggiamento, affinché prendano in animo le sorti del proprio destino senza attendere l'iniziativa di altri. Questa, cari colleghi, è la logica di uno Stato sociale fai da te e di chi dice «chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, scordammoce 'o passato».

mi sia concesso in premessa di esprimerle il mio pieno appoggio per la conduzione dei lavori. Non abbiamo compreso le critiche che le sono state prima rivolte dal collega Barbolini, anzi, apprezziamo la benevolenza che mostra nella gestione dei lavori di quest'Aula. Quindi, rigettiamo le critiche che le sono state in precedenza

Grazie,

con un sostanziale inutilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, con un effetto di taglio delle risorse destinate alle infrastrutture e, quindi, di blocco del credito d'imposta per gli investimenti nelle Regioni meridionali. meridionali. Inoltre il DPEF prevede, in vista della ripresa economica del 2010, il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati, allo scopo di ridurre Grazie,

coesione. Conferma l'obiettivo programmatico di destinare parte della spesa complessiva nazionale in conto capitale al Mezzogiorno e di continuare il processo di riequilibrio delle dotazioni di infrastrutture dell'area. Conserva la piena operatività degli strumenti di incentivazione, quali il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta potenziata dal ripristino dei tetti finanziari e dai controlli amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione.

come l'anno scorso, è positivo per il Nord, Nord che è la locomotiva economica per tutto il Paese, locomotiva che non può essere spenta ma va alimentata meglio: deve essere lasciata libera di crescere. Concludendo,

numeri presentati nel DPEF per dimostrare due gravi difetti della politica economica del Governo, un difetto di verità nei confronti del Paese nel presentare e presentare e perciò interpretare la natura della crisi e un grave difetto di coraggio nel predisporre le misure necessarie per affrontare la crisi. Sulla prima questione, il Ministro questa mattina ha detto che aveva previsto tutto.

risposto che la crisi non c'era e che eravamo dei disfattisti. Poi avevate detto che la crisi era di natura psicologica, poi che la crisi era solo finanziaria e non avrebbe avuto conseguenze sull'economia reale, poi che la crisi c'era ma per l'Italia non era molto grave, grave, poi che la crisi c'era stata ma non c'era più. Arriva il momento della verità e nel DPEF dovete scrivere e riconoscere

un punto in più di quanto avevate stimato solo tre mesi fa. Ancora nel settembre dell'anno scorso, quando la crisi aveva dimostrato tutta la sua terribile estensione, pensavate di poter proporre una crescita dello 0,5

Perciò, signori della maggioranza, si riscontra un grave difetto di verità che ha ritardato l'assunzione di responsabilità, perché purtroppo la crisi non è passata. Ci auguriamo che i timidi segnali di ripresa nel lontano Est si trasferiscano anche all'economia occidentale. Ci auguriamo che una possibile, ulteriore crisi del sistema delle carte di credito non esponga

per centinaia di migliaia di famiglie che perdono il loro reddito, per centinaia di migliaia di artigiani, di piccoli commercianti, di professionisti, di lavoratori precari che saranno espulsi dal sistema produttivo. Per affrontare questa stagione così difficile non c'è nulla, e qui si viene alla seconda questione: cosa fa il Governo?

gli stessi soldi, sempre quelli e sempre pochi e comunque che non escono mai delle casse dello Stato, per presentare un piano straordinario di interventi. Qui sarebbe interessante fare la storia, anche se purtroppo non ne il tempo e dunque mi Nel DPEF si dice che finalmente si attiva il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Bene, è una storia molto interessante perché si tratta dei denari che erano già stati stanziati in appositi fondi

dormito per qualche altro mese e finalmente sono poi stati restituiti alla destinazione assegnata loro dal Governo Prodi, solo che nel frattempo erano passati due anni e in mezzo era intervenuto il più grave razionamento creditizio nella recente storia economica italiana per le imprese. Il Governo aveva i soldi ed è rimasto a guardare. In secondo luogo, la sorda lotta di potere che attraversa il PdL siciliano (perché di questo si tratta) obbliga il Governo a promettere 7 miliardi di euro come prima *tranche*

Abbiamo dimostrato che questi soldi, semplicemente, non ci sono perché il FAS è stato prosciugato per i più svariati interventi e il Mezzogiorno è così rimasto senza presidio, nel cuore della più grave crisi economica.

dicono che, al colmo della più grave depressione dei consumi, il sostegno dato ai redditi è pari allo 0,17 del PIL. A quelli che stanno fuori dal circuito lavorativo (che sono i più poveri dei poveri, perché non hanno neanche potuto perdere il lavoro perché non lo avevano) voi dedicato lo 0,01 per cento,

realizzazione pressoché pari a zero, come dimostrano i dati dell'Associazione nazionale costruttori, mentre il dato del DPEF è quello vero. In quella tabella voi

0,6 punti in più rispetto all'anno precedente. Almeno, dovete chiedere scusa al Governo Prodi per gli insulti che gli avete rivolto. In conclusione, questi dati svelano una verità semplice: voi avete rinunciato ad agire, scegliendo di aspettare che passi la tempesta. Però, di fronte alla grandine, le famiglie e le imprese sono senza ombrello e senza rete antigrandine. nulla per una vigorosa difesa anticongiunturale. Non vi è nessuna ambizione riformista. Vi ha difettato il coraggio di dire la verità al Paese. Vi ha difettato la tempra di un coraggio riformista. però, ci sarebbe bisogno della visione lungimirante dello statista e non del buon venditore; del coraggio di proporre mete difficili e ambiziose. Avreste i voti per farlo, ma vi difetta il coraggio. Nell'immortale aria del "Don Giovanni" di Mozart si canta: «Vorrei e non vorrei. Mi trema un poco il cor». Quelle, però, erano pene d'amore e a uno statista non è consentito che tremi Amici e colleghi lombardi, come ricorda il grande lombardo don Lisander Manzoni, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. Ma chi coraggio non ha, non può governare bene una Nazione.

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare l'atto d'indirizzo che accompagna il Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2010-2013 proposto dal Governo e, a sentire i colleghi dell'opposizione, staremmo per deliberare su un documento puramente formale. Il concetto, infatti, da essi espresso ormai è costante: il DPEF non affronta le questioni strutturali economiche e sociali, non indica le prospettive per lo sviluppo dell'economia, non contiene una strategia di finanza pubblica. Quasi a voler legittimare l'idea che il Governo non sia in grado di guidare la crisi e sia solo alla ricerca del consenso. Un concetto espresso più o meno in questi termini dall'onorevole Bersani qualche giorni fa alla Camera dei deputati e che adesso lei riprende, senatore Giaretta. Mentre, invece a noi, al contrario, sembra che il Governo sia ben consapevole della fase che stiamo attraversando e degli strumenti da utilizzare per venire fuori da una difficile situazione. Lo testimoniano le dichiarazioni del ministro Tremonti nel corso delle audizioni che, meglio di ogni altro commento, hanno riassunto l'atteggiamento e le intenzioni dell'Esecutivo: cogliere, cioè, l'opportunità di trasformare l'attuale crisi in un'occasione di rilancio dell'economia italiana e di un più generale progresso del Paese. Il Governo quindi non nasconde (e come potrebbe farlo?) gli andamenti negativi di aggregati e i saldi di finanza pubblica: disavanzo, spesa primaria, fabbisogno, debito, tutte grandezze ulteriormente peggiorate in quest'ultimo anno, come ricordato e ripetuto da tutti coloro che sono intervenuti nel corso della discussione, anche se una lettura più attenta potrebbe mettere sotto una luce diversa questi stessi dati. Solo per memoria, ricordo a tutti noi la differenza tra andamenti nominali e strutturali dei saldi, quelli cioè depurati dall'impatto della congiuntura economica e, tenendo conto che l'impatto è valutato nel 2009 in un meno 2,2 per cento, l'indebitamento netto per l'anno in corso, ad esempio, non non sarebbe del 5,3 per cento sul PIL, ma del 3,1, come correttamente ha segnalato nella sua relazione il governatore Draghi, anche se qualcuno si ostina a fingere di non sentirlo. Ed il sensibile scarto per il 2009 si registra anche nelle annualità successive. Certo, un'informazione più articolata aiuterebbe ad alleviare la fatale polemica tra maggioranza ed opposizione condotta all'insegna della sterile logica «o tutto o niente». Andamenti negativi peggiorati nel corso di questo anno, dicevo, che però hanno una storia lunga e sono frutto anche delle dissennate politiche del Governo Prodi. E allora come non ricordare, come faceva giustamente il presidente Baldassarri in questa Aula,

Come non rimanere dubbiosi sul cosiddetto risanamento attuato dal ministro Padoa-Schioppa con i mancati pagamenti, quelli di cui tante imprese si lamentano? E lo scalone, senatore Giaretta, non lo abbiamo tolto noi;

Come non ricordare poi gli automatismi della spesa di enti locali e di sanità e il loro deficit fuori controllo, Regioni sulle quali voi dovreste fare delle approfondite riflessioni? E dove sono finiti i 18 miliardi di tesoretto amministrati o,

Colleghi, per cortesia. È l'ultimo intervento, poi si vota. Chi non è interessato alle dichiarazioni di voto può uscire dall'Aula. Prego, senatrice Bonfrisco. BONFRISCO *(PdL)*. Grazie, Presidente. Dicevo, la recessione non è finita ed il Governo non indugia a tranquillizzanti quanto irresponsabili dichiarazioni su una prossima ripresa né ammicca ai pur presenti aspetti positivi che il senatore Morando si è premurato di ricordarci. E' da questa consapevolezza complessiva che il Governo parte per impostare una nuova manovra economica e finanziaria volta ad accompagnare l'Italia fuori dalla crisi, prima, e a sostenerne la ripresa economica, poi. Innanzitutto rafforzando i pilastri che, dall'autunno 2008 - quel DPEF del 2008! -, ne hanno sostenuto l'azione: il supporto all'economia, la tutela del risparmio e del sistema creditizio, la salvaguardia della coesione sociale come fattore economico e non solo sociale. Basti pensare alle misure contenute nel recente decreto-legge n. 78, approvato dalla Camera, che continuano nel solco del sostegno delle famiglie e dell'occupazione e del rilancio degli investimenti delle imprese. Oppure all'indispensabile disposizione, senatore Lusi, che nell'assestamento ha consentito di sbloccare residui passivi per oltre 18 miliardi di euro, dovuti ai mancati pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Vorrei qui ricordare che l'insieme delle misure a tutela del risparmio e del sistema creditizio, a sostegno di redditi e consumi, per gli ammortizzatori sociali, varate dal Parlamento tra la fine del 2008 e l'inizio di questo anno, insieme all'assestamento del bilancio 2009 e al decreto-legge anticrisi ora in discussione qui in Senato, costituiscono un intero pacchetto di interventi anticongiunturali che vale circa 3 punti di PIL, oltre 50 miliardi di euro negli anni della programmazione davanti a noi. Altro che i pannicelli caldi evocati dal partito de «la Repubblica» di qualche giorno fa! Quindi, prevedendo rilevanti investimenti, umani e materiali, pubblici e privati, per il recupero della produttività e la crescita economica. Le finalità di sostegno alla crescita e recupero di produttività sono garantite anche dalla graduale realizzazione delle necessarie riforme mai sufficienti in questo Paese - dell'assetto istituzionale ed amministrativo in corso, come quella della pubblica amministrazione o che dovranno essere impiantate e sviluppate, come quella relativa al federalismo fiscale o alle pensioni. Una serie di iniziative, peraltro, che non devono e non possono essere valutate unicamente in relazione all'ammontare delle risorse finanziarie impiegate, ma anche agli effetti indiretti che esse avranno sul sistema economico, in termini di semplificazione, di sburocratizzazione e di rinnovata mentalità. Il tutto in un quadro di stabilità dei conti pubblici, un bene primario irrinunciabile, costituzionale. Questo è l'aspetto che giustamente preoccupa di più il Governo e conferisce alla sua azione, sino dall'emanazione del decreto-legge n. 112 del 2008, il senso del rigore, sinonimo in questo caso di prudenza, senatore Morando, e non di rassegnazione o addirittura di paura. Non possiamo dimenticare che il problema cruciale della nostra economia è il debito pubblico, il suo peso e la sua sostenibilità, oggi e per il futuro. Ce lo ha ricordato bene anche il Governatore della Banca d'Italia («L'elevato peso del debito rappresenterà una delle eredità più gravi della crisi») e ce lo ricorda il DPEF, che prevede una crescita del rapporto con il PIL fino al 2011, dove raggiunge il 118 per cento, per poi ridiscendere. Ovvio, quindi, che decisioni di spesa in termini anticiclici debbano essere considerate con particolare cautela. Ovvio, perché alla spalle c'è un'impostazione differente, una ricetta diversa e più impegnativa di quella del "tassa e spendi". Siamo sicuri, senatore Morando, che in questo momento fare debito - perché di questo si tratterebbe, con l'invito che ormai ci rivolgete da tempo - e trasferirlo alle prossime generazioni abbia un impatto così positivo sul sistema delle aspettative? Per l'attuazione del piano programmatico il Governo è impegnato in una sorta di difficile quadratura del cerchio tra uscite per le finalità di cui sopra, necessità di trovare risorse senza operare un rialzo della pressione fiscale e garantire la sostenibilità della finanza pubblica nel medio e nel lungo periodo. Un'operazione che si basa sul contenimento della spesa, specialmente quella corrente primaria, e sul rafforzamento del contrasto all'evasione;

con un incremento dell'8 per cento rispetto al 2007. Questi sono i dati ricordati nella recente relazione in materia. Tale aspetto, senatore Barbolini, rimarca il diverso approccio di cultura economica

volta al controllo del disavanzo pubblico e ha l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, sebbene rinviato di un anno, che ha riscosso l'apprezzamento delle istituzioni europee nel marzo scorso, in sede di aggiornamento del Patto di stabilità, e di istituzioni internazionali, compreso il Fondo monetario internazionale. Ricordo solamente che l'OCSE, poco più di un mese fa, ha definito molto saggio l'approccio del Governo nel definire le azioni per fronteggiare la crisi, a partire dalle misure introdotte anche a seguito delle decisioni assunte in sede europea già dal settembre 2008. Quella predisposta dall'Esecutivo appare quindi una manovra realistica e selettiva, consapevole cioè che non è possibile fare tutto e subito: dalla riduzione della spesa a quella della pressione fiscale, dalle riforme alle privatizzazioni. È un po' di tempo, colleghi dell'opposizione, che si è chiusa l'epoca dell'utopia, quella che tanto vi era cara: «siamo realisti, vogliamo l'impossibile». È questa una manovra su cui il Governo e la maggioranza che lo sostiene non si sottraggono da alcun confronto, consapevoli che tutto può essere oggetto di critiche, ma quelle legittime sono diverse da quelle preconcette. Da ultimo, il voto che convintamente il Gruppo del Popolo della Libertà esprime a favore della proposta di risoluzione firmata dai senatori Gasparri e Bricolo è forse legato al fatto che questo DPEF

il DPEF è finalizzato a consentire al Parlamento di conoscere con congruo anticipo le linee di politica economica e finanziaria del Governo. Ma a differenza di una norma, costituisce una dichiarazione di intenti, che non presenta una sanzione se non quella politica. È per questa ragione che presenta carenze nel rapporto tra la parte analitica e quella propositiva. Quindi, i rilievi fatti dai colleghi, anche dell'opposizione, sulle insufficienze del documento di oggi in esame riguardano le insufficienze strutturali e l'ottimismo a volte disarmante che accompagnano da oltre 20 anni lo strumento in sé: quella sorta di libro dei sogni, come prima giustamente è stato definito come è stato definito anche da noi, che non rimpiangeremo quando entrerà in vigore uno strumento più consono a una nuova stagione programmatoria, come quello previsto nel provvedimento di riforma della contabilità pubblica già approvato dal Senato. Anche in virtù di questo, il nostro voto è convintamente favorevole.

discutere. Stiamo affrontando temi molto importanti che riguardano il nostro Paese e proprio per queste ragioni - come lei ben sa - nella Conferenza dei Capigruppo svoltasi la settimana scorsa,

come a tutti i senatori, per averlo appreso dalla stampa, la presenza del Ministro ad una conferenza stampa. Siccome riteniamo sia assolutamente indispensabile che il signor Ministro sia questo pomeriggio in Aula a dibattere insieme a noi, anche perché apprendiamo

Senatore Giambrone, al momento la Presidenza ha avuto conferma che il ministro Bondi sarà presente in Aula.

Mi sarebbe piaciuto però avere il Ministro, perché è lui ad aver fatto delle dichiarazioni sul Fondo unico per lo spettacolo, non il Sottosegretario.

altresì il Sottosegretario che era presente prima. Non avevo alcuna intenzione di offenderlo, anche se ho visto che la sua reazione è stata piuttosto stizzita, ma mi sembrava che, data la rilevanza dell'argomento, la presenza del Ministro

Signor Ministro, colleghi, vorrei iniziare questo mio intervento riprendendo uno *slogan* che è stato molto spesso usato in questi tempi: se la cultura è un costo, pensate l'ignoranza. Eppure la cultura dovrebbe pacificamente essere considerata un valore aggiunto per ogni civiltà, un investimento e non un costo, non un lusso, ma un bene prezioso per ogni Paese. Peraltro, in Italia la cultura è anche una risorsa economica importante del nostro PIL e quindi uno strumento per contrastare la crisi in atto. Ecco perché, signor Ministro, non ci spieghiamo quali siano le ragioni dei tagli apportati al Fondo unico per lo spettacolo,

Il Fondo unico per lo spettacolo, lo sappiamo tutti, è nato nel 1985 e prevede una serie di interventi, in una sorta di regolamentazione unitaria, a favore di enti, istituzioni, associazioni che si occupano di teatro, cinematografia, musica, danza e così finanziamenti, dipende la vita e l'attività di molti teatri, ma anche di produzioni cinematografiche che si avvalgono di questi contributi statali e delle associazioni di cultura che fanno attività sul territorio.

Il ministro Bondi - ecco il motivo dell'importanza della sua presenza - aveva recentemente promesso un reintegro del Fondo unico per lo spettacolo.

prevedere nei prossimi provvedimenti di finanza pubblica una modalità per reintegrare questo Fondo. Dico che non è bastato perché anche oggi abbiamo letto sulla stampa che il presidente Berlusconi ha intenzione di varare nuovi provvedimenti in materia finanziaria per rivedere alcune disposizioni del decreto anticrisi, ma del Fondo unico per lo spettacolo non si parla. È evidente che la

ripeto, in modo provocatorio - questa domanda: il teatro può vivere senza soldi pubblici? Egli si è dato anche una risposta positiva, ma è evidente che la sua è stata una provocazione,

sarebbe difficile pensare ad una sopravvivenza di questo modo di fare cultura senza soldi pubblici. È evidente però che può capitare che i costi di produzione di questo tipo di spettacoli possano aumentare in presenza di contributi pubblici, dal momento che questi possono generare (e sottolineo possono) comportamenti impropri da parte degli amministratori. Inoltre, una terza criticità che si può verificare con questo tipo di normativa oggi vigente è rappresentata dal fatto che i sussidi pubblici possono creare anche artificialmente un'offerta culturale per la quale non esiste domanda. Quindi, signor Ministro, anche se non è questo l'oggetto delle mozioni oggi in esame, la invito a ripensare ad un sistema di finanziamento del mondo dello spettacolo e della cultura, nell'attuale situazione normativa dobbiamo assolutamente pensare che un sostegno pubblico ci debba essere.

possano trovare presto una pronta soluzione, perché credo che il nostro Paese e la nostra civiltà meritino che la cultura sia collocata al primo posto e riceva grande attenzione da parte dei Governi, di qualsiasi colore essi siano.

colleghe e colleghi, finalmente si può parlare di cultura in quest'Aula, perché è precisamente dall'ottobre scorso che chiediamo che se ne parli, avendo presentato una mozione già a quell'epoca. Purtroppo, arriviamo a parlarne in una condizione di grande emergenza, o meglio di allarme (perché di vero e proprio allarme si tratta). L'hanno denunciato in molti, come abbiamo fatto anche noi parlamentari (di opposizione, ma anche di maggioranza),

in molti abbiamo denunciato questo problema ed ha espresso la propria viva preoccupazione il Presidente della Repubblica, che ha sinceramente auspicato che si ponga dignitosamente rimedio ad una situazione che personalmente trovo paradossale, oltre che miope e difficilmente comprensibile a chi ci guarda dall'estero, magari persino con un punta di comprensibile invidia. Il Paese con la maggior densità di beni culturali e con il più grande patrimonio in termini di creatività e tradizione musicale, teatrale e cinematografica lascia morire ed esaurire lentamente questa ricchezza, anziché valorizzarla: siamo davvero un Paese bizzarro, signor Ministro. Ma veniamo ai fatti, che sono esposti nella nostra mozione:

un intervento che insieme al *tax credit* per il cinema aveva dato al settore nell'immediato un po' di respiro e per il futuro garanzie di risorse e riforme.

teatri, teatri di tradizione, compagnie di danza e cinema, per non parlare delle fondazioni lirico-musicali. Chiudono? Non ci importa - risponde il Governo - e non ci interessa nemmeno che siano a rischio circa 250.000 posti di lavoro e chiudano tante piccole imprese collegate con la produzione culturale. Si fa meno cinema? Non c'è problema.

hanno protestato vivacemente. Sono arrivati anche a minacciare di boicottare la più importante manifestazione cinematografica del nostro Paese: la Mostra del cinema di Venezia. Come si può restare indifferenti a questo grido di dolore? dolore? In quest'Aula non dovrebbe essere certo necessario ricordare che quando parliamo di attività come il teatro e il cinema parliamo di industria culturale, di impresa e creatività insieme, una potenzialità esplosiva se la si sa coltivare con intelligenza e lungimiranza, anziché lasciarla agonizzare. Un esempio di vitalità possibile viene dai dati di «Roma economia» del 2006-2007, secondo i quali il settore cinematografico conta già oltre mille imprese attive direttamente nella produzione e distribuzione e nelle attività radiotelevisive. Invece, la spesa pubblica per la cultura nel nostro Paese costituisce meno dello 0,3 per cento del bilancio. Che cos'è rispetto al 2 o al 3 per cento dei Paesi più competitivi? Voglio fare ancora l'esempio del cinema di cui stiamo discutendo in 7a Commissione del Senato, forse anche con eccessiva lentezza. FUS (quest'anno circa 71 milioni di euro) si deve finanziare tutta la filiera: la produzione, la distribuzione, l'esercizio, la promozione, la formazione, l'attività delle istituzioni e degli enti cinematografici pubblici. un niente. Per avere un termine di paragone con quanto avviene invece in altri Stati d'Europa, posso fare ancora una volta l'esempio del Francia, dove il Centro nazionale per la cinematografia, che - com'è noto - è un ente pubblico di gestione di tutti gli interventi di sostegno e promozione, ha a disposizione più di 525 milioni di euro. E il presidente Sarkozy, che non è certo di sinistra, ha aumentato i fondi per la cultura nel suo complesso. Quindi, siamo davvero molto indietro rispetto all'assunzione della cultura come fattore di sviluppo, come una delle molle che acquistano sempre più centralità nella strategia complessiva di sviluppo di un Paese moderno che sa vedere il nuovo, quel nuovo di cui parla Jeremy Rifkin: il fatto cioè che la cultura è sempre più un canale privilegiato di produzione di pensiero innovativo e di sollecitazione all'innovazione, un potente «veicolo e generatore d'innovazione e sviluppo». Ma dobbiamo davvero arrivare a pensare, colleghi della maggioranza, che sia vera la generalizzazione secondo la quale, quando governa la destra, la cultura non solo non viene considerata fattore di sviluppo civile ed economico, ma viene soffocata in tutte le sue espressioni? Infatti, questo è già questo il tema della mozione n. 173, ma non si può non richiamare anche la sofferenza di altre istituzioni qualificanti della nostra identità culturale e storica, come le biblioteche nazionali e pubbliche e gli archivi di Stato che non riescono più nemmeno a garantire un orario di apertura decente. Per non parlare delle istituzioni culturali che rappresentano un prezioso patrimonio archivistico e documentale, che fanno ricerca e formazione di prima grandezza e che quest'anno hanno subito, anche loro, una decurtazione di più di 2 milioni di euro. Alcune di esse, molto prestigiose, che finora hanno rappresentato anche simbolicamente la nostra identità civica e culturale sono rimaste escluse dai finanziamenti pubblici. Voglio citarne qui soltanto alcune; di fondazioni legate ai nomi di Pascoli, D'Annunzio, Vico, Mazzini e Matteotti: niente più dal pubblico prenderanno da qui in avanti, è una storia cancellata.

di introdurre misure più efficaci. La risposta, mi dispiace ricordarglielo, è stata il silenzio, anzi la connivenza con il ministro Tremonti. Logica vorrebbe, signor Ministro - non lo dico in chiave

un gesto forte ma che forse servirebbe a segnalare l'inopportunità di una riduzione di risorse di questa portata, che atterra e azzera i nostri istituti culturali.

ai colleghi, che questo ramo del Parlamento, che in tanti momenti attraverso la Commissione di merito ha saputo esprimere posizioni comuni sulla cultura, voglia farlo anche in questa occasione. *(Applausi

come noto il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163. La finalità, precisata all'articolo 1 della suddetta legge, è quella del sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni ed iniziative di rilevanza nazionale da svolgere in Italia e all'estero. Come stabilito dall'articolo 15 della citata legge n. 163 del 1985, al finanziamento del FUS si provvede ogni anno mediante la legge finanziaria. Le somme stanziate per il FUS sono indicate in tale legge nella Tabella C, distinte per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio. Dato che si tratta di trasferimenti di spese correnti sono impegnabili unicamente gli stanziamenti del primo anno e dunque gli stanziamenti per il secondo e terzo anno

Il riparto della somma disponibile per il 2009 è stato così stabilito dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2009: 47,5 per cento agli enti lirici, 18,5 per cento alle attività cinematografiche, 16,3 per cento alle attività di prosa,

L'industria dello spettacolo è di estrema importanza per la vita del nostro Paese. Come evidenzia la ponderosa relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo dell'anno 2007 (l'ultima relazione disponibile), le imprese coinvolte sono numerose: per la produzione cinematografica, gli stabilimenti e le imprese di produzione, le imprese di sviluppo e stampa, le imprese di doppiaggio, le imprese di distribuzione e noleggio, gli esercizi cinematografici esclusivi o polivalenti; per la musica, gli enti autonomi lirici e sinfonici, cioè le fondazioni (14 le maggiori in Italia), le imprese liriche, le imprese concertistiche, le imprese di spettacolo e di balletto, le imprese di spettacolo di operette, i complessi orchestrali di musica leggera, i complessi bandistici; per il teatro, i teatri stabili, le compagnie di prosa, le compagnie di rivista e varietà, le compagnie di commedia musicale, gli esercizi teatrali; per i trattenimenti vari, gli spettacoli viaggianti, i circhi equestri, le imprese organizzatrici di festival. Nel 2007 sono state presentate ben 5.187 domande di sovvenzione al Fondo e i beneficiari sono stati 2.948, di cui: 14 fondazioni lirico sinfoniche, 1.075 imprese nel settore della musica, 135 in quello della danza, 422 in quello della prosa, 73 in quello dei circhi, 56 in quello dello spettacolo viaggiante, 1.173 in quello del cinema. Gli incentivi del FUS impattano, quindi, su una vasta platea di imprese, per la cui vita economica sono spesso assai determinanti. La grande rilevanza economica dell'azione del FUS è meglio compresa se si tiene conto dell'importanza del numero degli addetti, qui ricordato dalla senatrice Franco, che è di Molti di questi addetti hanno professionalità di estremo rilievo, anche internazionale: sono vere bandiere dell'Italia nel mondo.

Ma come sappiamo bene, il mondo dello spettacolo, parte assai rilevante dell'industria culturale nazionale, è di estrema importanza per la stessa identità ed immagine del nostro Paese, non solo in Italia ma anche all'estero. un solo esempio, l'opera lirica, che è stata per secoli una delle principali modalità di apprendimento della lingua italiana all'estero, è tuttora un formidabile veicolo di comunicazione della nostra identità culturale. L'opera lirica e la musica sinfonica costituiscono ricchezze culturali e patrimoni identitari del nostro Paese e sono ancora oggi uno dei prodotti culturali di eccellenza, che meglio rappresentano nel mondo il *made in Italy*. La piena consapevolezza dell'importanza del ruolo del FUS nella nostra economia e vita sociale, brevemente riassunta nelle precedenti considerazioni, è alla base della mozione n. 178 del PdL che sto illustrando. La richiesta principale fatta al Governo nella nostra mozione è di uno stanziamento integrativo straordinario nel Fondo unico per lo spettacolo per il corrente esercizio finanziario, che riporti le disponibilità a livello di quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Siamo convinti che il mancato reintegro del Fondo provocherebbe gravi ripercussioni, anche occupazionali, in settori di attività del nostro Paese di importanza strategica, in particolare nella presente situazione di crisi. La mozione si sofferma sulla forte criticità della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, alle quali è destinata un'aliquota del FUS di poco inferiore al 50 per cento. Per esse, l'impegno richiesto al Governo, contestualmente al reintegro del finanziamento del è quello di provvedere a una riforma sistemica, in linea con i contenuti di una risoluzione approvata in 7a Commissione il 18 marzo scorso su un apposito affare assegnato. Tale riforma dovrà puntare sia a una diversa *governance* delle fondazioni, che responsabilizzi meglio gli amministratori e li stimoli a operare secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio, sia a promuovere una maggiore presenza di finanziatori privati incentivati da apposite facilitazioni fiscali. Ricordo che la risoluzione approvata in Commissione (il documento XXIV, n. 3) conteneva vari impegni per il Governo, tra cui quelli volti a garantire un aumento significativo delle risorse da destinarsi al FUS; prevedere specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; destinare una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; incentivare un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; introdurre adeguate misure volte ad accrescere la produttività del settore; richiedere alle fondazioni lirico-sinfoniche che gli statuti attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero al sovraintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché un'adeguata autonomia decisionale; mettere in campo ogni azione volta ad incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, garantendo agevolazioni fiscali alla contribuzione privata; privata; valorizzare le finalità e il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo presso i giovani, la loro *mission* di trasmissione di valori civili fondamentali verso cui, del resto, sono sempre state orientale le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. Più in generale, la mozione impegna il Governo ad avviare una riforma complessiva dei meccanismi di finanziamento delle attività di spettacolo che tenga conto degli indici effettivi di affluenza del pubblico, di resa aziendale e di efficienza gestionale, nonché della quantità e qualità della proposta culturale. In sostanza, si chiede l'instaurazione di nuove modalità di finanziamento che siano premiali rispetto all'effettivo apprezzamento da parte del pubblico fruitore e alla correttezza dell'azione amministrativa dei gestori. signor Ministro, chiediamo al Governo un pronto ripensamento su questo finanziamento.

non ripeterò quanto è stato già detto su cui, peraltro, c'è una condivisione di fondo e una comunanza di vedute, come emerge chiaramente dalle mozioni che sono state presentate. Mi permetto, però, di fare qualche breve osservazione di carattere generale.

La ragione è molto semplice: evitare finanziamenti a pioggia, parziali, articolati in mille rivoli che in ogni legge finanziaria venivano inseriti a seconda

che doveva obbedire ad una serie di regole di carattere generale e che avrebbe potuto incentivare e sostenere tutte le forme di manifestazioni culturali, dello spettacolo in genere, che avessero una funzione importante sotto il profilo sociale,

il compito, di anno in anno, ferme restando le regole generali ed astratte e i criteri per il finanziamento, di reperire e definire la dotazione annua di questo Fondo in ragione della programmazione che, nell'ambito del mondo della cultura, ogni anno si effettuava e del fabbisogno e delle esigenze che in questo settore emergevano.

il meccanismo delle manovre economiche

un valore marginale: si interviene con manovre estive o con altri interventi e, nell'ambito di questi, si applicano dei correttivi, si interviene sul piano economico e finanziario. Ed è quello che è successo e sta succedendo con riferimento al al finanziamento del FUS. Questo però ha un'altra ripercussione, dal nostro punto di vista estremamente negativa, cioè salta il meccanismo della programmazione. Un conto infatti è che vi sia la certezza di un sistema di regole generali che si applicano a tutti,

individua le risorse, certo nei limiti della compatibilità generale di bilancio, un'altro conto è che nel primo trimestre, a metà anno o nel terzo trimestre, a prescindere dalla legge finanziaria, intervenga un decreto che, per ragioni ovviamente legate ai vincoli di finanza pubblica, comincia ad introdurre una serie di tagli, più o meno lineari, che colpiscono i vari settori e quindi mettono in crisi la programmazione del Ministero. Questo è il punto. Questo è l'elemento di crisi. Ora, questo è avvenuto.

scritto che si trova di fronte ad una situazione di contrazione delle risorse pubbliche che certamente inciderà sull'eliminazione di alcuni sprechi (se ve ne sono, e certamente ve ne saranno), ma che, a regime e nel corso dell'attività di programmazione, colpisce una serie di attività importanti: il Ministro citava il caso della Mostra del cinema di Venezia, della Scala di Milano, dell'Arena di Verona, del San Carlo di Napoli e del Maggio fiorentino, che non possono essere annoverati tra coloro i quali sono destinatari dell'"elemosina pubblica", come per la verità è stata definita oggi dal Presidente del Consiglio, il quale ha preannunziato che venerdì in Consiglio dei ministri si varerà un decreto-legge con cui si rimpinguerà il FUS. Noi dobbiamo intervenire su questo È chiaro però che per farlo c'è bisogna di un sistema e di una dinamica di programmazione economica e finanziaria che non mettano a rischio la continuità dell'attività amministrativa e di programmazione, soprattutto quando questa, nel settore della cultura, è una variabile indipendente rispetto alla ordinarietà dell'attività amministrativa che si fa nei vari settori dell'amministrazione dello Stato e delle Regioni. La cultura non è equiparabile ad altri settori e non può subire un taglio lineare senza che questo incida immediatamente sulla creazione del prodotto culturale, sulla sua possibilità di essere veicolato a livello nazionale e internazionale e quant'altro.

perché è giusto anche quello che si dice rispetto alla circostanza che nel momento in cui non vi è il controllo dei meccanismi di spesa, l'assenza di razionalizzazione determina una serie di *enclave*, di privilegi che poi mettono a rischio la credibilità dell'intero sistema di finanziamento alla cultura. Il dato di fondo, però, con esso dobbiamo fare i conti e di questo devono assumersi la responsabilità il Governo e noi tutti, Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. Se mi è consentito, c'è un solo errore che non possiamo e non dobbiamo fare:

essere travolte dal conformismo della regola del mercato. Già ormai la regola del mercato non funziona più dove dovrebbe funzionare per ragioni che non sta a noi qui approfondire e se noi immaginassimo di fare una riforma che abbia come sola impostazione la circostanza che i finanziamenti si danno solo ed esclusivamente a quelle attività che fanno cassa, poiché purtroppo il livello di crescita culturale del nostro Paese ha modelli diversi, non tutti compatibili o ascrivibili alle logiche

su richiesta delle Commissioni riunite 5a e 6a, al fine di consentire un approfondito esame del decreto-legge anticrisi, la seduta dell'Assemblea prevista per domani pomeriggio non avrà luogo. Inoltre, previ accordi intercorsi tra i Gruppi, informo l'Assemblea che la replica del Governo sulle mozioni in discussione, nonché le dichiarazioni di voto e il voto finale sono rinviati a venerdì mattina, alle ore 9. Informo altresì che domani, alle ore 12, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l'aggiornamento del calendario dei lavori.

Onorevole Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, qualche tempo fa, in occasione della dichiarazione di voto sulla mozione per la promozione della cultura, ho avuto modo di sottolineare la grande attenzione che da sempre la Lega Nord pone alla cultura del territorio, radicata nelle tradizioni popolari, nelle lingue locali, in usi e costumi e in ogni espressione artistica, a partire dai repertori teatrali, musicali e letterari. Non a caso, ci battiamo contro lo Stato centralista che, per forza di cose, tende a omologare un territorio che, nel caso della nostra penisola, custodisce qualcosa come il 60 per cento di tutte le opere d'arte mondiali. Far finta di nulla e consentire l'omogeneizzazione di un simile patrimonio sarebbe, dal nostro punto di vista, un vero e proprio affronto alla cultura. Con il federalismo siamo tesi al recupero del vissuto identitario dei popoli da cui discendiamo; un patrimonio da non disperdere in tempi di globalizzazione e massificazione culturale estrema, tendente all'annullamento dell'identità, quando invece è proprio un'identità forte a consentire la sopravvivenza culturale, oltre che economica. La cultura umanistica e la letteratura locale sono puntualmente oggetto di promozione, memorizzazione e divulgazione da parte delle nostre amministrazioni, attraverso biblioteche e scuole. Azioni simili vengono svolte per la musica, le arti figurative e lo spettacolo in genere. Nel contesto attuale, caratterizzato dalla drastica riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, che tra sprechi, privilegi, rendite di posizione e assistenzialismo non ha dato sempre buona prova di sé, emerge però l'attività delle Regioni, che si è sempre più sviluppata negli anni, pur in assenza di una legislazione statale di cornice, prevedendo investimenti sul piano della progettazione, della promozione, della comunicazione e del sostegno alle diverse iniziative culturali del territorio. In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, molte Regioni hanno provveduto al riordino della propria legislazione in materia di spettacolo ispirandosi a principi comuni, quali l'affermazione del valore sociale ed economico dell'attività, l'approccio integrato alla materia, il ricorso a modalità di sostegno economico differenziate, tali da prevedere sia contributi finanziari, sia incentivazioni sul piano economico e fiscale. Al di là, quindi, degli interventi ai quali si sta lavorando per ridare ossigeno al settore (estensione dello statuto delle piccole e medie imprese a quelle dello spettacolo, accesso al credito agevolato, stimolo allo sviluppo attraverso la defiscalizzazione degli investimenti, strumenti a difesa dell'occupazione e ammortizzatori sociali), appare quanto mai necessario, oltre al recupero urgente delle somme tagliate, che mettono a rischio migliaia di imprese e relativi posti di lavoro, un ripensamento dell'attuale sistema di gestione ed erogazione dei finanziamenti pubblici allo spettacolo, assicurando a questi continuità, tempestività e congruenza, superando il carattere nazionale del FUS e restituendo alle Regioni la loro fondamentale importanza nel settore. Chiediamo in pratica una riforma organica del sistema di gestione e distribuzione dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo che si ispiri ad un modello di gestione che riconosca alle Regioni un ruolo più incisivo, anche attraverso il coordinamento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attribuendo poteri di gestione diretta dei fondi da parte delle Regioni per i profili per i quali, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004, non occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale.

evidenza un disagio che non è dell'opposizione politica o di un partito, ma purtroppo di una gran parte dell'opinione pubblica italiana e straniera: come, infatti, si può giudicare un taglio di 200 milioni di risorse, sui 544 complessivi grazie all'integrazione dell'ultimo Governo Prodi, quando l'Italia è conosciuta nel mondo anche e soprattutto per la sua arte millenaria, per la sua cultura musicale, e lirica in particolare, per il suo cinema, con gli Oscar e i premi ottenuti ovunque? 7a Commissione, addirittura, attraverso il presidente Possa, su richiesta dei colleghi Vita e Giambrone, ha affrontato un affare assegnato sui tagli consistenti agli enti lirici, ha ascoltato i direttori della Scala, delle fondazioni liriche di Napoli, di Roma e di Verona, ha approvato - il ministro Bondi lo sa bene - una risoluzione unanime con un suo parere favorevole che aveva promesso il ristabilimento immediato di quei fondi. Ieri abbiamo parlato del DPEF, abbiamo parlato in molti e purtroppo non abbastanza dei tagli alla cultura, dei tagli ai saperi. Ci siamo posti, signor Ministro, una domanda: se quelle alla cultura, se quelle in particolare per lo spettacolo fossero risorse per i costi o per gli investimenti, quando le nostre opere liriche sono rappresentate nei teatri di Tokyo e Shanghai, ed è l'Italia in quel momento ad essere rappresentata nel mondo, quando attraverso il cinema italiano candidato agli Oscar è l'eccellenza italiana, è l'Italia di cui noi tutti, centro, destra o sinistra, dobbiamo essere orgogliosi, come può la 7a Commissione discutere in questo momento della nuova legge *bipartisan* sullo spettacolo dal vivo con un taglio del 40 per cento delle risorse?

in particolare alle fondazioni culturali storiche, come la «Giacomo Matteotti» e come la «Giovanni Pascoli». Il sottosegretario Giro è intervenuto sempre in terza persona, parlando del Governo come un fatto a lui estraneo, come se un destino cinico e baro fosse contrario a queste fondazioni così meritevoli. Lo dico, signor Ministro, perché è un altro argomento su cui vorremmo sentire la sua parola,

proposito delle battute infelici sugli insegnanti e le prove di dialetto, per ricordare loro che, ad esempio, Carlo Porta con le sue opere appartiene alla cultura italiana a pieno titolo

mi auguro sia solo un collegamento infelice, il mio - le prove di dialetto della Lega non andrebbero male con le dimenticanze e i ritardi del Governo nei preparativi per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

Si possono approvare le mozioni, ma si debbono trovare risorse vere: le promesse sono state troppe. L'Italia non può essere declassata alla serie B anche nello spettacolo e il Governo e lei, Ministro, non potete esserne responsabili.

Qui ci vorrebbe un altro Fondo per lo spettacolo per concentrare in cinque minuti quello che uno ha da dire! Ho aggiunto la mia firma alla mozione presentata dal senatore Possa ed altri e, caro Ministro, lei ha un compito formidabile e noi vogliamo esserle di sostegno. È assolutamente indispensabile che si ricostituiscano questi fondi e lei, siamo certi, si batterà in prima linea perché ciò avvenga. Infatti, se ad un cospicuo fondo andiamo a tagliare una quota si creano problemi, ma si assorbe la botta; se ad un fondo già assai modesto si apporta un taglio, si rischia il tracollo. quindi assolutamente necessario, come qualcuno ha detto più felicemente di me, che si metta bensì in cantiere una riforma, ma stando attenti a non arrivare a luci della ribalta spente. quindi intervenire assolutamente, tenuto presente che i magri fondi che tutti i Governi (sottolineo tutti), da decenni a questa parte - e purtroppo comincio ad averne non breve memoria - hanno destinato a questo settore, debbano essere assolutamente confermati o rimpolpati. Naturalmente, con premialità per gli enti virtuosi, perché molto si è sprecato. Che vogliamo negare? Ormai lo hanno riconosciuto anche autorevoli operatori dello spettacolo e personaggi che hanno da dir la loro, anche in termini di esperienza. Si è parlato della lirica e certo è un capitolo fondamentale, ma le potrei dire, signor Ministro, che non ci sono solo i grandi enti. Potrei dire, per esperienza diretta, che il teatro lirico sperimentale "Adriano Belli", che licenzia da decenni i principali cantanti dai propri concorsi, che poi diventano le grandi *star*, si arrabatta con poche decine di migliaia di euro, risparmiando su un mazzo di cantinelle o su dieci costumi per mettere in piedi la propria rassegna

quindi il vero problema: non soltanto puntare su poche istituzioni, ma cercare di arrivare a ciò che produce realmente in questo settore.

che hanno dilapidato a volte in spettacoli insignificanti o culturalmente negativi gran parte di quel poco che avevano a disposizione e la gente ha pagato. Non c'è dubbio che anche in questo settore l'apporto e la sinergia del privato sono indispensabili, c'è poco da fare. Potremmo dire, con una formula superficiale ma significativa, che l'apporto pubblico è fondamentale e imprescindibile, ma certo non risolverà da solo i problemi. Bisogna trovare le formule, le sintesi, le affascinanti sintesi, che pure sono percorribili, perché si possa riattrarre del capitale per investimento privato in questo settore, come accade in molti altri Paesi del mondo. Vorrei dire anche, all'interno di questo grande capitolo, che noi sottolineiamo la scarsezza di risorse per la lirica o anche per alcuni settori della musica, per non parlare della danza, ma dimentichiamo che l'Italia ha grandi tradizioni ed enormi potenzialità nel teatro di prosa. E se vado a vedere, nell'ambito della miseria sulla quale ci dibattiamo da decenni, devo rilevare che abbiamo un 16,3 per cento delle risorse destinate alla prosa che mi sembra, nella lotta tra poveri, essere assolutamente inaccettabile. Certo, che si prenda come unico indice quello dell'afflusso di spettatori agli spettacoli è uno *slogan* suggestivo, ma insidioso; è certamente ora di finirla con gli spettacoli finanziati col denaro pubblico privi di spettatori, perché questa è un'indecenza a cui abbiamo assistito per troppo tempo, ma, nello stesso tempo, poiché lo scadimento del gusto e l'orientamento del gusto stesso è un'altra realtà dura da affrontare, da affrontare, bisogna tener conto di molti elementi, tra i quali questo, ma che non sia l'unico indice. In conclusione, bisogna dare assolutamente ascolto al grido di dolore che viene oggi da questo mondo. Dobbiamo fare ogni sforzo, come maggioranza di Governo ma anche come intero ceto politico, per dare un segno preciso e concreto, non di qui a qualche anno, quando la riforma prenderà corpo, ma immediatamente. Concludo col dire che in questa materia è giusto intervenire, ma è giusto farlo quel tanto che necessita, perché il mondo dell'arte e della creatività non debbono essere ingabbiati da una legislazione troppo stringente. Dobbiamo dare sostegno nel senso di creare, più che leggi, un clima di comprensione e di sostegno al mondo della creatività artistica. Questo è il suo grande compito, onorevole Ministro, più che leggi, norme e codicilli, perché l'arte dev'essere libera e lo spettacolo deve godere della sua libertà creativa. Quindi, a noi creare le coordinate legislative di sostegno perché abbia libero campo tale creatività.

colleghe e colleghi senatori, signor Ministro, sono molto grata al mio Gruppo per aver presentato la mozione n. 173, dandoci in questo modo la possibilità di portare all'interno di quest'Aula il grido di dolore e l'allarme che il mondo dello spettacolo italiano sta lanciando dai diversi territori del Paese. In questi giorni non c'è grande manifestazione dalla quale non si levi la richiesta di aiuto contro i tagli al Fondo unico per lo spettacolo. Per noi si tratta dì continuare il discorso intrapreso con una precedente risoluzione sulla cultura, presentata dalla collega Sbarbati, perché appunto la lirica, il teatro, il cinema, la danza e l'attività circense fanno parte del più ampio mondo della cultura, quel mondo che purtroppo in questa fase della politica italiana è assolutamente ai margini dei pensieri come anche degli interventi del Governo. Già durante l'approvazione della finanziaria 2009 il Partito Democratico ha tentato in tutti i modi di opporsi al taglio del FUS per riportarlo al livello della finanziaria Prodi del 2007, con la quale si è cercato almeno di ripristinare in parte i fondi drasticamente ridotti dal precedente Governo Berlusconi. Questa nostra battaglia non era e non è una battaglia ideologica di salvaguardia di pochi interessi particolari e, voglio ribadirlo, non è nemmeno la difesa di un settore che ingiustamente qualcuno della maggioranza tenta strumentalmente di far rientrare nell'alveo politico della sinistra. Salvaguardare il mondo dello spettacolo non è di destra, né di sinistra, ma è nell'interesse del Paese. Voler bene alle attività dello spettacolo vuol dire voler bene all'Italia, a quella straordinaria creatività che l'ha fatta grande nella storia e nel mondo. Pensiamo veramente di poter risolvere i problemi della grave crisi economica e della finanza pubblica tagliando i già minimi fondi del FUS? Sapete meglio di me che siamo uno dei Paesi in cui l'investimento pubblico per lo spettacolo è tra i più bassi e, nonostante ciò, riusciamo costantemente a produrre eccellenza in tutti i suoi comparti, ad organizzare eventi di grande risonanza. Sono convinta anch'io che tutto il sistema necessita di profonde riforme, che l'attuale legislazione va rivisitata, in accordo con le Regioni e con le autonomie locali; noi siamo disposti a fare la nostra parte, ma non possiamo aspettare una nuova legge, mentre tutto il sistema va a rotoli, Stiamo parlando di un settore con 250.000 addetti, con più di 6.000 imprese, che producono indotto, che arricchiscono l'offerta turistica, che promuovono i singoli territori. La messa in ginocchio di questo comparto significa la messa in ginocchio di un intero comparto produttivo, che non è sostenuto né da interventi anticrisi e nemmeno dagli ammortizzatori sociali. Anche dalla mia Regione, terra di confine e di cultura, è partito un coro di proteste contro il taglio al FUS; lo abbiamo sentito in alcune importanti manifestazioni, come il "Mittelfest" di Cividale e il premio cinematografico "Sergio Amidei" di Gorizia. Il futuro di otto teatri di prosa, del Lirico "Verdi" di Trieste, dei cinque festival cinematografici e di altre attività è strettamente legato ai finanziamenti statali e regionali. Ridimensionare questa ricca attività, che si è complessivamente caratterizzata negli ultimi anni anche per l'impegno nella costruzione di

e dell'integrazione linguistica e culturale come uno dei suoi aspetti di eccellenza, vorrebbe dire impoverire un intero territorio e la sua popolazione. un'ultima considerazione riguardante il Teatro stabile di lingua slovena di Trieste, che si trova in questo momento in una grave difficoltà finanziaria, perché oltre alla penalizzazione del FUS è stato anche penalizzato dai mancati contributi delle altre autonomie autonomie locali (Regione, Provincia e Comune). Mi sembra che - cito le parole del ministro Frattini di qualche giorno fa a Trieste - il rispetto delle specificità delle minoranze in questo ambito del teatro

credo che grida di dolore e cori di protesta siano tutti comprensibili e possono anche avere le loro ragioni, ma penso che in quest'Aula in tale occasione dobbiamo fare una riflessione, del tipo di quella proposta nel bell'intervento del senatore D'Alia e, a mio giudizio, anche dall'ottima mozione del senatore Possa, sui meccanismi istituzionali della finanza pubblica. Tutti Tutti ricordano questo Fondo istituito alla metà degli anni Ottanta e inserito nella finanziaria, ma nessuno ha avuto, almeno nei testi scritti, l'onestà intellettuale di ricordare

rifiutato prerogative e competenze sullo spettacolo, perché quando il Ministero per i beni culturali era nato il modello era un altro.

Bondi e Tremonti come se fossero due sindacalisti. No, devo dire che anche nelle grandi difficoltà io ho apprezzato il ministro Bondi, perché ha onorato l'idea del Governo come organo collegiale, nel quale non esistono posizioni individuali. Quando esistono, non si fa più parte del Governo. Per questo, mi sono sembrate ingenerose le considerazioni della senatrice Franco, più pertinenti ma a mio giudizio erronee, perché ella si è richiamata alla Francia. Ma la

per vent'anni non è mai stata inserita in nessuno dei meccanismi previsti dalle misure anticrisi assunte dai vari Governi? Se vogliamo questa concezione della cultura, allora non possiamo il ministro Bondi nel suo rapporto con il Governo di cui fa parte. Evidentemente, c'è un problema di dislocazione istituzionale diversa e questo va al di là dell'emergenza, da cui mi auguro si possa uscire grazie anche a questo dibattito. PRESIDENTE.

signor Ministro per la sua presenza costante durante questo dibattito. È da ormai quasi un anno che l'opposizione ha richiamato il Governo, il Parlamento ed il Paese sui rischi che i tagli inferti al FUS arrecano al complesso del sistema culturale italiano. Parto dall'ultimo intervento, quello dell'amico senatore Compagna. Non credo che si possa riformare qualcosa che muore per asfissia. Credo che tutte le legittime proposte di riforma verranno apprezzate e discusse, ci si confronterà e probabilmente ci sarà anche una forte dialettica su questo signor Ministro lo sa, noi siamo sempre stati disponibili al confronto nella 7a Commissione, però ritengo che, prima di riformare, bisogna salvare. E oggi siamo in condizioni di difficoltà addirittura per il mantenimento in vita. La consapevolezza che la riduzione di oltre 70 milioni di euro comporta l'inevitabile messa in mora per i teatri, per il cinema, per la musica classica e lirica è affiorata prepotentemente nell'opinione pubblica. Non è solo uno schiaffo all'identità del Paese, con tante buone tradizioni ed eccellenze nei più svariati settori, ma anche un colpo ferale inferto al sistema economico e produttivo di una grande e storica importanza. Stiamo infatti procedendo inevitabilmente alla dichiarazione della resa di un comparto che conta circa 6.000 imprese, 270.000 addetti, un distretto importante per il Paese e per le sue prospettive: il nostro cinema, i nostri autori di teatro, le tante compagnie di danza, la musica classica, quella lirica, tanta parte della storia d'Italia, della nostra storia di tradizione e di merito che oggi mettiamo in ginocchio con conseguenze inimmaginabili. Da qualche mese molti colleghi, anche della maggioranza, hanno avvertito questo tipo di grave rischio, e insieme stiamo portando avanti un'istanza comune per la salvezza della nostra cultura; poi lavoreremo per l'eventuale ristrutturazione, rivisitazione, ricomprensione e rilancio della stessa. Gli incontri con il Presidente della Repubblica, con il Presidente della Camera e con il Presidente del Senato hanno voluto significare questa grande attenzione da parte di tutti. Nonostante i tentativi fatti in questi anni, anche di risanamento, i nostri enti lirici versano in grave difficoltà e il nostro cinema è al collasso. Il senso di questa disfatta viene reso benissimo da una cifra: la cultura in Italia vale meno dello 0,2 del PIL. Mai così poco da tanti decenni. La cultura è vissuta - ahimè, ormai possiamo dirlo con certezza - come un costo da questo Governo nella sua collegialità, e lo sottolineo perché so che il ministro Bondi si sta battendo per reperire fondi. In realtà la cultura non è un costo: la cultura deve essere un investimento. Questo Governo ha un'idea di cos'è lo spettacolo? Sa come procedere nel campo delle riforme? Oppure si pensa che il taglio del FUS sarà funzionale ad un sistema culturale con una nuova era, che magari avrà solo due fondazioni lirico-sinfoniche, qualche film (pochi, probabilmente) e la liquidazione del teatro, della danza e di tante alte attività? Se è questo il modello, si dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Non credo, signor Ministro, che si voglia questo. La Francia forse non è un riferimento, ma lo è sicuramente per l'entità degli investimenti fatti fatti e credo si possa dire che è anche un esempio. In questi giorni numerose e condivisibili sono le polemiche in corso sulla scarsa attenzione che il Governo sta dimostrando anche riguardo alle celebrazioni dell'Unità d'Italia: il primo finanziamento pubblico dello spettacolo in Italia risale al 1861, signor Ministro, data dell'Unità d'Italia, e fu firmato dal presidente Cavour poco prima della sua morte; era rivolto in particolare al Teatro Regio di Torino. I finanziamenti attuali sono dunque frutto di una tradizione che ha 150 anni e che tanti capolavori ha prodotto in tutti i settori, rendendo gli italiani più consapevoli, ricchi e apprezzati nel mondo.

finanziando teatri, auditorium, sale e infrastrutture culturali. Non è un'esagerazione: se il FUS non venisse immediatamente riportato almeno a 460 milioni di euro e la stessa cifra non fosse confermata per il 2010, le conseguenze sarebbero evidenti a tutti. Molte delle 13 istituzioni lirico-sinfoniche italiane dovrebbero chiudere per fallimento, molte tra le *tournée* delle compagnie teatrali sarebbero annullate, metà dei 280.000 lavoratori dello spettacolo resterebbe senza lavoro e la produzione cinematografica entrerebbe in una crisi che non ha precedenti. Se la sentono i colleghi della maggioranza e del Governo ed il Ministro qua presente di legare i loro nomi a questa tragedia annunciata? Credo di no, anche perché ritengo che l'impegno ci sia.

Signora Presidente, signor Ministro, in questi giorni abbiamo assistito a manifestazioni polemiche e attacchi, in parte anche comprensibili, contro il ridimensionamento del Fondo unico per lo spettacolo. Abbiamo ascoltato con il consueto rispetto il richiamo del Capo dello Stato come le preoccupazioni dei rappresentanti dei lavoratori. È indubbio che la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo attuata dal Governo rappresenti un danno per un settore importante per l'economia italiana un appannamento dell'immagine stessa del Paese, che da sempre beneficia dei teatri, della lirica, della genialità dei direttori d'orchestra come della professionalità di scenografi e costumisti. La dotazione del FUS è stata ridotta da 500 milioni nel 2003 sino a 398 milioni nel 2009. È ovvio che gli stanziamenti per la cultura risentano del ciclo economico: è più facile trovare risorse quando il PIL non subisce una contrazione di più del per cento. È drammaticamente scontato che in questo momento critico si debba tener sotto controllo il debito pubblico e trovare le risorse per sostenere i redditi di quanti hanno perso o stanno perdendo il posto di lavoro. Il punto però è che, a mio avviso, è stata considerata in modo poco adeguato la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo che, se mantenuta, provocherebbe una serie di crisi occupazionali. Non sarebbe solo un danno alla cultura, all'immagine e alla storia stessa del nostro Paese, ma potrebbe aggravare la crisi economica mettendo in difficoltà ben 200.000 lavoratori Inoltre, è sicuramente ancora presente nella politica ed in parte anche nella società civile un pregiudizio, cioè considerare la spesa in cultura come improduttiva, quasi uno spreco. Non è così. E disinvestire oggi in questo settore significherebbe danneggiare anche uno dei principali punti di attrazione del nostro Paese per il turismo internazionale. Certo, non possiamo neanche nasconderci dietro un dito e gridare allo scandalo senza affrontare le riforme. Il FUS è uno strumento arcaico, figlio anche di logiche meramente assistenziali, e se c'è una parte dell'offerta culturale che deve essere sostenuta, anche se in perdita, esiste un enorme patrimonio che può camminare con le proprie gambe,

Dobbiamo cioè evitare finanziamenti a pioggia, selezionando in base a precisi criteri meritocratici i progetti da finanziare e quelli da abbandonare. Come falliscono le imprese inefficienti possono fallire anche i teatri. Quello però che non possiamo fare è ridurre drasticamente il FUS nel giro di un anno e far fallire la metà dei teatri, grandi e piccoli. Questa non sarebbe una razionalizzazione e nemmeno una riforma, ma solo un errore strategico, un passo indietro potenzialmente letale per il mondo dello spettacolo. La soluzione è accelerare i diversi progetti di riforma che il Parlamento sta discutendo. Faccio alcuni esempi: la VII Commissione della Camera dei deputati sta discutendo una proposta di legge sullo spettacolo dal vivo che prevede di assegnare nuove funzioni alla Conferenza unificata, mettendola in condizione di programmare nel triennio gli interventi e i finanziamenti, di promuovere accordi e scambi internazionali e, soprattutto, di semplificare e snellire tutte le autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli. Il testo del progetto di legge mira inoltre a favorire la fusione tra società, associazioni ed enti culturali, anche appartenenti a settori diversi, per renderli economicamente più solidi, e a rifondare completamente il sistema di sussidio pubblico, favorendo l'esenzione delle imposte sugli avanzi di gestione reinvestiti per per ammodernare i teatri. La riforma delle attività cinematografiche (già avviata in Senato in un clima di grande condivisione) prevede la nascita di un Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, attraverso il quale unificare competenze amministrative e gestionali attualmente sparpagliate ed opache, oltre all'istituzione di un nuovo canale di finanziamento per il settore che avrebbe il notevole pregio di non gravare sul bilancio dello Stato. Nel settore del cinema il mercato ha già attuato autonomamente la diminuzione del 20 per cento degli investimenti pubblici è stata infatti già compensata dall'aumento del 30 per cento degli investimenti da parte dei privati. L'occupazione è raddoppiata e la quota di mercato dei film italiani è risalita fino al 30 per cento. Questa *partnership* tra pubblico e privato può essere il modello da seguire in tutto il settore della cultura e dello spettacolo. I talenti di certo non mancheranno: almeno su questo non ci sono dubbi. Per completezza, cito infine la riforma già annunciata da lei, signor Ministro, delle fondazioni lirico-sinfoniche, che speriamo di discutere presto in quest'Aula. Noi siamo con lei e

cercano, anche in modo molto coeso, di aiutarla a fare qualcosa per la nostra cultura.

Tuttavia, prima di affrontare brevemente la nostra rimostranza per la mancanza di rappresentanza all'interno del Consiglio di Presidenza

Non so se sono state prese decisioni in assenza della nostra componente politica. So per certo che se l'Italia dei Valori fosse stata rappresentata

Segnalo altresì che, in merito alle problematiche da me sollevate in altre occasioni (in sede di discussione del bilancio interno del Senato) in relazione alla assegnazione degli appalti all'interno dell'amministrazione, nonché alla composizione delle commissioni di gara non ho ricevuto ad oggi alcuna risposta.

(che doveva esserci dal primo giorno di questa legislatura) all'interno del Consiglio di Presidenza per controllare e verificare circostanze che a noi oggi restano oscure. L'oscurità assoluta è questa impossibilità di dire no,

aggiunge che siamo consapevoli del problema; se ne discute spesso in Conferenza dei Capigruppo e il Presidente stesso si è fatto promotore di varie proposte,

Grazie, Presidente. un pianto della Magna Grecia. Quasi tutti i parlamentari del Meridione si sono infatti lamentati per come stanno procedendo i finanziamenti per il Mezzogiorno. Devo però riportare che i giornali di oggi e i telegiornali di ieri hanno parlato dell'ospedale di Agrigento.